disponibilità nel visionare una risposta all'interrogazione del collega Palma sui possibili beneficiari della norma contenuta nella finanziaria in relazione ai reati amministrativi. Posso accettare, anche se non la condivido, l'idea che un sindacato ispettivo venga limitato nei suoi contenuti; quello che non posso invece accettare è che nell'atto, che è in disponibilità di visione in Commissione, vi siano pagine intere di nominativi che non sono presenti per il fatto che si fa riferimento agli *omissis*

Se la Corte dei conti ha trasmesso un documento che rappresenta oggettivamente una dimostrazione di omertà di Stato (perché vengono cancellati, in un atto destinato al Parlamento, dei nominativi su semplice richiesta dell'interessato), mi chiedo se il Governo non intenda rappresentare che la Corte dei conti, nel

poliambulatori che hanno convenzione diretta con il Parlamento della Repubblica.

con trasporto via elicottero fino ad Avezzano, evidentemente se ci sono dei problemi gravi per quanto riguarda i colleghi - senza voler intervenire su nessuno, però

Pensavo avesse terminato, prego. CASTELLI *(LNP)*. Forse dovrebbe stare più attento, perché avevo appena finito di dire che intendevo sviluppare il ragionamento nei termini previsti dal Regolamento. Allora, se mi consente, signor Presidente, siccome non è la prima volta che mi toglie la parola senza averne diritto,

addivenire prima all'esame del successivo provvedimento di legge previsto nella seduta odierna, per un motivo che adesso andrò a spiegare. Anch'io sono rimasto molto colpito dalle parole del collega Gramazio nel suo intervento stamattina, quando ha denunciato una serie di questioni assai rilevanti per il Lazio, da

ma ritengo sia necessario approfondire anche questo tema. D'altro canto, stiamo erogando una serie assolutamente importante di fondi per migliorare la sanità, in

Regolamento del Senato, il Gruppo di cui mi onoro di essere Presidente fa proprio il disegno di legge n. 1509, comunicato alla Presidenza il 18 aprile 2007, recante il titolo: «Modifica della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente

proprio per l'aspettativa che ha creato nella stampa, sui quotidiani, nei *media* e quindi nell'opinione pubblica, dovrebbe essere affrontato con la massima celerità. Per tali motivi, si chiede l'inversione giorno. Alcuni aspetti, all'interno di questo disegno di legge, comportano la mia adesione alla proposta del senatore Castelli e vanno considerati in maniera assolutamente prioritaria. Spesso si dice che la Costituzione non non è più in aderenza con i tempi o si parla di norme che devono regolare il dettato costituzionale per giungere a dei rapporti sociali e civili, come quelli in questione, adatti al tempo ed agli anni in cui viviamo, ma altrettanto spesso non si interviene con la dovuta celerità e con la dovuta attenzione. Proprio

la quale affonda le proprie radici nel diritto di famiglia romanistica e di una tramontata potestà maritale, non più coerente con i princìpi dell'ordinamento e con il valore costituzionale dell'eguaglianza tra uomo e donna».

la conversione di un decreto-legge o è data dalla necessità di tranquillizzare gli amministratori che devono far quadrare i conti con quel provvedimento, grazie alla conversione di quel decreto‑legge, dopo che li hanno già fatti mezzi quadrare, intervenendo con delle poste di bilancio in attesa della conversione del decreto-legge che è in corso di discussione? Da un lato,

una questione che nei nostri cittadini è profondamente e fortemente radicata come coscienza sociale, civile e storica.

Mi colpisce che su un provvedimento tanto importante, che interessa milioni di famiglie italiane, la Lega faccia ostruzionismo

di approvare molto più in là il provvedimento in modo che le famiglie italiane continuino a pagare ancora per un po' i 10 euro di *ticket*, rifiutando un'azione stringente e bersagliando questo provvedimento.

il Governo, il ministro Turco in particolare, per la sensibilità che ha maturato nel corso del dibattito parlamentare. Diversi di noi, anche nel precedente passaggio al Senato, di fronte alla proposta positiva del Governo di ridurre il *ticket* da 10 a 3,5 euro - un passaggio importante - avevano insistito su come quella misura, il mantenimento cioè dei 3,5 euro, fosse di fatto anacronistica. Non solo continuava ad essere un'ingiustizia per molte famiglie italiane, ma si pensava e si calcolava che il costo dell'esenzione di quella quota di *ticket* fosse maggiore rispetto ai vantaggi che il bilancio pubblico ne potesse avere. Il primo passaggio al Senato è stato complicato. Vi erano problemi di copertura. Diversi di noi come il sottoscritto hanno presentato un emendamento per l'eliminazione totale del *ticket*. Abbiamo discusso

una copertura più precisa ci hanno permesso di cogliere il frutto di una iniziativa parlamentare ampia e forte.

i parlamentari del centro-sinistra hanno dato questo contributo di analisi al Governo ed hanno saputo cogliere con particolare attenzione un tema così importante per la salute e la vita di milioni di famiglie italiane.

prevede un intervento straordinario dello Stato per ripianare il *deficit* sanitario di alcune Regioni e già la natura del provvedimento, per come è impostato e per le finalità che si propone, non può che lasciare molte perplessità e tanti dubbi. Il principio dell'autonomia, della separazione, quel federalismo strisciante al quale ci siamo più volte riferiti sembra capovolto completamente e sembra essere ritornata quella che una volta si diceva essere la politica della privatizzazione degli utili e della pubblicizzazione delle perdite. Ma, al di là delle considerazioni di ordine generale e facendo riferimento agli interventi che mi hanno preceduto, in modo particolare a quelli dei senatori Cursi e Gramazio che mi trovano assolutamente concorde, voglio sottolineare un aspetto fondamentale delle finalità di questa legge che soccorre Regioni che hanno dimostrato di non avere la capacità di gestire una sanità sana,

l'emergenza rifiuti e l'emergenza sanità, tra parentesi tra di esse strettamente collegate sicché l'emergenza rifiuti ha provocato una sorta di aumento esponenziale di patologie tumorali e di altre malattie. Ma riferendoci solo a quella sanitaria, signor Presidente, non posso non rilevare come la gestione della sanità in Campania sia stata fallimentare.

nel momento in cui si pone a capo di un'intera politica sanitaria di una Regione un dirigente che non ha dato sicuramente buona prova di sé, si dà il segnale si dà il segnale della gestione di una sanità politica, non di una politica sanitaria, vale a dire una gestione scandalosa, clientelare, che non riesce a soddisfare le esigenze minime in un campo così delicato come quello della salute e della tutela della sicurezza. quella gestione clientelare ha fatto sì che la gestione sanitaria diventasse anche gestione politica, gestione sul territorio, gestione delle liste, degli inserimenti a livello delle consulenze e dei più biechi favoritismi, tant'è che il *deficit* della Regione Campania è uno è uno dei maggiori e dei più allarmanti. Se questa è la sanità in Campania, se la Campania è la Regione in cui si compiono statisticamente più viaggi della speranza verso altre Regioni che sicuramente hanno un modello se la gestione della sanità in Campania deve essere aiutata nel momento in cui ha creato essa stessa tali deficienze e tali condizioni, non vedo la necessità per cui bisogna prestare soccorso per perpetuare un sistema, un'organizzazione, una deriva istituzionale e politica che potrebbe essere poi avvantaggiata anche da strumenti finanziari così importanti. Più volte la Regione Campania ha tentato di appianare il debito, più volte quelle programmazioni

aumentare le sue capacità politiche di inserirsi in un sistema che diventa una sorta di grimaldello antidemocratico perché altera gli equilibri sul territorio, ebbene non posso che essere

che appunto si sta per ultimare - «può proporre che venga richiesto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro». Faccio questa richiesta, signor Presidente, perché, alla luce degli interventi di oggi, la determinazione di questa Camera non può prescindere da informazioni più dettagliate in merito al

Il senatore Tomassini con il suo intervento mi ha dato modo di verificare l'opportunità di ricorrere all'articolo 98

Senatore Franco, la richiesta di parere del CNEL rappresenta - secondo il parere espresso il 23 ottobre 2001 dalla Giunta per il Regolamento una variante specifica di questione sospensiva e pertanto deve essere avanzata prima dell'inizio della discussione generale. Essa può essere ammessa anche nel corso della discussione generale solo a fronte di nuovi elementi emersi nel corso del dibattito.

il dibattito che si è svolto in quest'Aula, così come la discussione che si è svolta in Commissione. Vorrei che ritornassimo sul tema, perché qui si è svolta una discussione di carattere più generale sulle modalità di gestione e sulle linee di politica sanitaria in questo Paese, che forse potrà svolgersi in modo più utile in altra sede. Rispetto alle questioni sollevate, ritengo che ci troviamo di fronte ad un provvedimento che, nei fatti, è un provvedimento di attuazione della legge finanziaria, perché c'è un contesto. Quindi, quando ci si solleva il problema anche del coordinamento tra le diverse responsabilità istituzionali e il nodo del coordinamento tra le diverse responsabilità istituzionali,

Il fondo transitorio - mi dispiace dover fare una lezione, ma devo parlare dei contenuti e del merito del provvedimento, mentre qui spesso si è parlato d'altro - nasce infatti con la legge finanziaria, nasce con lo stanziamento di un milione di euro. Questo provvedimento, il cui fondo peraltro - lo dico anche rispetto alle obiezioni che sono state sollevate in ordine al coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni

e Province autonome di Trento e di Bolzano, che ne hanno espresso la condivisione. Quindi, rispetto agli argomenti che sono stati sollevati, mi sembra non ci siano i presupposti per tenere la discussione su questo livello. Vorrei anche precisare che il tavolo tecnico di verifica per gli adempimenti risale all'intesa del 23 marzo 2005, quindi certamente non ad un provvedimento che è stato inventato oggi. Il problema vero è quello della responsabilità che questo Governo si è assunto in ordine alla questione dei disavanzi relativi ad esercizi pregressi per la gestione della sanità, un problema che non è nato né nel 2006 e nemmeno nel periodo immediatamente antecedente e che è stato affrontato nel passato senza mai essere risolto. C'è invece qui un'assunzione di responsabilità del Governo, in coordinamento con i diversi livelli istituzionali, per superare definitivamente il tema, la questione e il nodo dei disavanzi pregressi in sanità, adottando piani concordati sui quali c'è un impegno, anche del Governo. Governo. La finalità, nel momento del risanamento, è infatti anche quella di garantire quel diritto che qui ho sentito evocare in molti interventi: il diritto costituzionalmente tutelato, non solo come diritto individuale, alla salute, ma anche come interesse generale della collettività. consenso ad un provvedimento che interviene in alcune Regioni con la finalità, da un lato, di superare una situazione deficitaria su cui maturano interessi (situazione che quindi è destinata a peggiorare), e, dall'altro, anche di assicurare alla cittadinanza per il presente e per il futuro

che qui è stata evocata (quella di un comportamento contraddittorio in ordine ai *ticket* e alla loro abrogazione), che questa è una discussione che resta agli atti parlamentari. Se ne è discusso nel contesto della manovra finanziaria e anche successivamente con la modifica delle proroghe. In Commissione Igiene e sanità, abbiamo approvato a maggioranza, fin dai tempi del documento di politica economica e finanziaria, un parere che prevedeva il finanziamento della sanità attraverso la fiscalità generale e progressiva. Il provvedimento oggi in discussione porta a compimento un impegno politico che il Governo si era assunto legge finanziaria; lo porta a compimento in anticipo, con un passaggio del Senato che ha trovato poi compimento alla Camera. Credo sia un provvedimento sul quale tutti dovremmo convenire.

Auspico davvero che questo giudizio di iniquità, che è arrivato da parte delle opposizioni, possa vederci consenzienti nel condurre con la stessa determinazione la medesima battaglia anche in quelle Regioni dove il *ticket* sulla diagnostica a 46 euro preesisteva all'introduzione che è stata fatta in finanziaria e potrebbe continuare a permanere anche dopo che lo avremo abrogato come *ticket* aggiuntivo per le altre Regioni.

dell'attuale sistema sanitario e quindi compromettano il diritto alla salute. È un provvedimento esecutivo della finanziaria - l'ha già ricordato la senatrice Emprin Gilardini - che introduce una novità: l'affiancamento dello Stato alle Regioni, i piani di rientro, con strumenti certi di responsabilizzazione delle Regioni. Non c'è pertanto alcuna compiacenza agli sprechi che sono stati giustamente condannati: Governo, Corte dei conti e, con l'emendamento di cui discutiamo dopo l'approvazione alla Camera, anche il Parlamento con le sue Commissioni dovranno vigilare corretta applicazione. Questi fondi vanno a coprire il pregresso e non possono in nessun caso essere utilizzati per la spesa corrente. Ovviamente il dimensionamento e la ripartizione interregionale del finanziamento nell'ambito del sistema sanitario sono legati ai LEA,

per ribadire il diritto costituzionale all'omogeneità delle prestazioni che sarebbe reso non esigibile se non si intervenisse sui debiti pregressi. La seconda obiezione riguarda gli strumenti per il monitoraggio, i controlli e le sanzioni. Ebbene, gli strumenti sono quelli già previsti dalla legge, con momenti abbastanza significativi di intervento sul bilancio regionale, addirittura l'aumento automatico di aliquote, che ovviamente sarebbe molto grave perché sarebbe

conviene mettere in evidenza le novità e io credo che la vera novità di questo testo sia la totale eliminazione della compartecipazione sulla diagnostica, l'eliminazione cioè dei *ticket*, con una copertura - lo voglio dire senza enfasi - sostanzialmente corretta.

Vorrei dire, con un orgoglio di tutti, maggioranza e opposizione, che l'eliminazione dei *ticket* è un'iniziativa, salvata in quest'Aula del Senato, della quale tutti dovremmo essere fieri - lo diceva il senatore Mazzarello - perché è un provvedimento rivolto a tutte le donne e a tutti gli uomini del Paese, il che rende molto più importante il decreto pur importante che abbiamo esaminato.

e le finanze*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero ringraziare i relatori, la senatrice Emprin Gilardini ed il senatore Tecce, e tutti i senatori intervenuti nel dibattito per il contribuito che hanno voluto portare

e Regioni, in sede di Conferenza Stato‑Regioni, ed è in linea con i presupposti contenuti nel Patto per la salute sottoscritto lo scorso settembre. I relatori hanno posto l'accento sulle modifiche intervenute alla Camera sul testo originariamente licenziato dal Senato, significativamente sull'abolizione del *ticket* sulla soppressione della norma riguardante l'impignorabilità delle somme. Non mi soffermerò sul contenuto di queste norme, che sono state dibattute e sono note a tutti nell'Aula. Nel corso del dibattito alcuni interventi dei senatori dell'opposizione si sono soffermati sul carattere del provvedimento, che conterrebbe una disparità di trattamento delle Regioni. Vorrei sottolineare in questa sede che la disponibilità delle risorse da destinare al ripiano dei disavanzi è vincolata, come è stato sottolineato, all'attivazione di un processo virtuoso che prevede il concorso finanziario delle Regioni interessate e l'affiancamento delle stesse per la realizzazione del percorso di rientro dal debito. Come è stato riconosciuto anche dagli interventi dei senatori dell'opposizione, le norme di rientro sono cogenti e pongono vincoli seri per chi le deve attuare. Credo si possa dire che in questo modo si cerca di porre rimedio ad una situazione oggettivamente difficile e si punti ad affermare l'esercizio di un'azione più consapevole, incisiva e responsabile da parte delle Regioni e degli amministratori delle aziende sanitarie locali. Nel corso dell'*iter* e a conclusione dei lavori delle Commissioni congiunte sono state richieste al Governo assicurazioni sia in relazione alla copertura che al ripristino delle competenze dei fondi ai quali si è fatto ricorso per la copertura del provvedimento stesso. Questa richiesta è stata riformulata in Aula anche dai relatori. Voglio ribadire all'Assemblea del Senato l'assicurazione che il Governo provvederà a rispettare gli impegni presi e a dare loro attuazione non appena si concluderà l'assestamento del bilancio nel mese prossimo venturo.

si chiede di rafforzare l'azione di raccordo con la Conferenza Stato-Regioni che, per inciso, è l'organo con il quale è stata concordata l'intesa preventiva sul testo del provvedimento che esaminiamo. Per queste ragioni il Governo chiede al Senato un voto favorevole alla conversione del decreto.

più Governo del Ministro non so chi ci sia. Eppure il Ministro sta zitto, tace, non dice nulla, credo con poco rispetto per l'Assemblea, per il suo ruolo

sarei interessato a sapere cosa pensa il Ministro di questo provvedimento e se ne pensa qualcosa, a questo punto, visto che se ne è stato zitto con aria distratta.

poi nella finanziaria 2008 avanzate la proposta di dimezzarle, così riducete ogni anno le tasse. Se il *ticket* l'avete introdotto voi, non mi sembra un gran risultato averlo tolto su spinta dell'opposizione,

fondi alla famiglia e alla ricerca. Ripeto, non mi sembra una grande risultato. La maggioranza ha una visione quanto meno pittoresca dell'economia e dell'amministrazione pubblica. Voi parlate sempre di doveri e mai di diritti: che la sanità sia un diritto per tutte le famiglie italiane è assolutamente indiscutibile, però forse vi sfugge che se in una certa Regione ci sono sprechi degli amministratori o non vengono pagate le tasse in modo adeguato, c'è poi qualche altra famiglia in qualche altra Regione che paga per la propria sanità e anche per la sanità degli altri. Quindi un pochino più di serietà e di rispetto

sono volte a chiedere all'Aula di votare il non passaggio agli articoli per delle considerazioni che lo vedono anche se ragionare a favore del decreto per l'abolizione del *ticket*, per dei ragionamenti che riguardano la spalmatura sul territorio di questa ingente somma di risorse del Tesoro, pari a circa 5 miliardi di euro nel periodo, che, secondo la nostra interpretazione e secondo i ragionamenti che abbiamo svolto nella prima lettura e che sono stati svolti nell'altro ramo del Parlamento, comportano una sperequazione nel territorio nazionale; infatti, vanno a premiare le Regioni non virtuose, cioè quelle che hanno speso di più e si sono indebitate con un'attività contraria, per quello che abbiamo rilevato stamattina ma che non è stato votato dall'Aula,

che la correzione operata nell'altro ramo del Parlamento in ordine alla copertura finanziaria per l'abolizione del *ticket*,

dell'introduzione della disposizione che elimina il *ticket* per la fascia dianzi ricordata da alcuni colleghi,

Questo ragionamento è probabilmente plausibile dal punto di vista politico, ma non lo è dal punto di vista della legge di contabilità. Non solo, ma il fatto che non è plausibile dal punto di vista della legge di contabilità è stato rilevato dalla Commissione bilancio, perché ho capito la difficoltà dei colleghi in Commissione bilancio, ma in tale Commissione il il parere è stato espresso come un parere di contrarietà che, nella proposta dell'opposizione, era un parere di contrarietà ai sensi dell'articolo 81 e che con sofferenza i colleghi della Commissione bilancio hanno

delle norme di contabilità, che come sappiamo sono leggi rafforzate, cioè con una valenza superiore alla legislazione normale, alle disposizioni usuali, e tutto questo potremmo farlo in pochissimo tempo. La proposta di non passaggio agli articoli avanzata dal senatore Galli, quindi,

(in quanto noi ripetiamo la nostra proposta), ma per colpa vostra viene ad essere fortemente violato e vulnerato.

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario. Osserva, altresì, che gli esiti della verifica annuale dei piani di rientro, a differenza della relazione sul riscontro dell'estinzione dei debiti, non viene trasmessa al Parlamento. A fini informativi sarebbe opportuno che tali elementi venissero forniti regolarmente anche al Parlamento così come utile sarebbe la trasmissione tempestiva degli esiti del tavolo

sulle quali il parere è contrario».

si propone di introdurre una forte misura sanzionatoria per gli amministratori delle Regioni in disavanzo che, nei tre anni successivi al 2005, continuino a peggiorare la situazione di indebitamento nel settore sanitario.

Il parere del Governo

l'emendamento 1.2. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

1.4 è volto a specificare che l'avvio da parte della Corte dei conti di un eventuale giudizio di responsabilità amministrativa e contabile nei confronti delle Regioni in disavanzo, debba essere accompagnato dall'adozione delle conseguenti misure sanzionatorie anche a carattere Troppo spesso infatti votiamo leggi che coprono buchi realizzati da amministratori che poi tranquillamente escono da queste loro azioni senza nessun tipo di responsabilità personale. Quindi, una volta accertata per incapacità, per dolo o per altro, questo tipo di azione, ci deve essere anche una giusta conseguenza. Invito quindi i colleghi a votare a

il puntuale pagamento delle rate concordate nelle procedure transattive stipulate con i creditori. Si ricorda, infatti, che alcune delle Regioni interessate dal presente decreto hanno provveduto a stipulare apposite transazioni con i loro creditori, che in molti casi hanno a loro volta ceduto il credito transatto agli istituti bancari e finanziari. L'impossibilità per alcune Regioni di ottemperare a tali accordi transattivi rischia conseguentemente di porre i creditori in una situazione di grave difficoltà giuridica e finanziaria. Questa è una cosa che spesso si sottovaluta, dimenticando che questi debiti, che vengono creati da molte Regioni in campo sanitario, si tramutano anche in situazioni di non pagamento di fornitori privati normalissimi, che non hanno nessun interesse particolare nel giro amministrativo pubblico, che semplicemente non riescono più a recuperare i propri soldi. Siccome le Regioni però con molta facilità promettono il rientro di questi debiti o crediti (dipende dai punti di vista), quando ciò non viene mantenuto spesso sono le aziende normali che di per sé vivrebbero di vita propria, che creano ricchezza vera, che hanno occupazione e impegnano persone in maniera assolutamente libera rispetto agli ambienti pubblici - che alla fine pagano per l'incapacità gestionale

Tale sanzione è individuata nella riduzione automatica dei finanziamenti statali nell'anno successivo allo sfondamento, fino ad integrare le coperture del maggiore disavanzo. Ogni volta che adottiamo questi provvedimenti si spergiura, da parte della maggioranza di turno, che è l'ultima volta. Evidentemente poi non succede così, perché a distanza di poco tempo ci si ritrova esattamente nella stessa situazione.

ai cittadini della Lombardia, del Veneto e anche di altre parti d'Italia che hanno ben amministrato la cattiva amministrazione di gente come Bassolino. Questa è la verità vera! Avete capito o no? LNP).* Ci vuole una bella «faccia di tola» per stendere una cortina fumogena come quella che state stendendo.

stampa o dai fotografi, di un fotografo che potrebbe anche fotografare atti del Governo oppure della stessa Presidenza. È alle sue spalle alla sinistra, dove normalmente non sono autorizzati a stare fotografi.

naturalmente i colleghi hanno notato che sulla copertura di questo provvedimento la Commissione bilancio ha di nuovo espresso un parere contrario, seppur senza far ricorso all'articolo 81 della Costituzione. È evidente il perché: incredibilmente e inopinatamente il Governo ha riproposto in questa Aula esattamente la stessa copertura che, di fatto, di fatto, il Senato non aveva ritenuto possibile, perché contraria, sotto vari profili, alle norme di contabilità pubblica

Signor Presidente, di nuovo abbiamo all'esame un provvedimento che presenta profili veramente molto problematici per ciò che concerne l'articolo 81 della una tranquillizzante dichiarazione del Governo sull'esistenza delle cifre nei capitoli previsti e il di più intervenuto in questa Aula, meglio, nell'aula della Commissione. Nessuno dei profili di problematicità è stato risolto. È una copertura in conto capitale per spesa corrente con conseguente dequalificazione della spesa. È una copertura che potrebbe crearci dei problemi con l'Unione Europea, problemi che per il momento non si prospettano perché il Governo assume l'impegno di rimpinguare quei capitoli, ma è un impegno che non sappiamo se e quando potrà effettivamente essere Soprattutto, è una copertura con una gestione fuori bilancio. Quest'ultimo aspetto è unanimemente riconosciuto dai colleghi di maggioranza e di opposizione come un *vulnus* vero e proprio all'articolo 81 della Costituzione. Francamente non so come il Presidente della Repubblica potrà consentire la promulgazione di quel decreto con quella copertura che egli stesso in

copre in maniera puntuale la stessa spesa. Per vero, il Governo di sinistra si contraddistingue per quella famosissima trasmissione della nostra infanzia e giovinezza: «Meglio tardi che mai».

È tempo che la politica riprenda il governo dell'economia. È tempo che il nostro Governo sappia che si possono trovare risorse in ossequio anche al programma elettorale che abbiamo presentato. Io avevo individuato tagli ai finanziamenti alle scuole non pubbliche e tagli al

il mancato *ticket* comporterebbe. Anzitutto, ci mancherebbe che noi non fossimo d'accordo ad abbassare la pressione fiscale ai cittadini. Però, bisogna anche essere onesti intellettualmente, bisogna svelare un imbroglio perché io mi indigno quanto si è indignato il collega Stefani, che ne ha tutte le ragioni, quando ho sentito in quest'Aula sbandierare con grande euforia il fatto che si va a privilegiare, ad aiutare qualche categoria di contribuenti pensando che i soldi si trovino così, per strada o accantonati. Se mi consente un paradosso, signor Presidente, ogni cittadino italiano, in quanto soggetto ad imposta, è un contribuente. Ma ogni cittadino italiano è anche parte di questo Stato, come contribuente deve dare. Ma in questo caso si va a sgravare il cittadino come contribuente di 500 milioni

Si sia almeno corretti e non disonesti politicamente, come si sta facendo in quest'Aula, facendo passare queste norme come un provvedimento che aiuterà qualcuno perché quel qualcuno, che avrà 500 in più, sarà lo stesso che dovrà dare 3.000 allo Stato come debito debito che lo Stato in questo caso ha nei confronti di tutta la Nazione.

Ovviamente esprimo un parere negativo in quanto tutta la materia è stata ampiamente discussa in sede di Commissione bilancio in relazione alla copertura, con un dibattito molto ampio. Ribadisco pertanto quel parere contrario, che per altro già nel voto dell'emendamento

La richiesta è stata formulata alle ore 17, ma ora sono le ore 19,30. Prevedendo dichiarazioni di voto, non vorrei mai pensare - non sono così maligno che la Presidenza intenda sottoporre al voto dell'Assemblea tale richiesta una volta concluso il provvedimento al nostro esame, perché voglio ricordare che questa

per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario», in scadenza il 19 maggio prossimo. È indispensabile dunque arrivare alla sua attesa approvazione a seguito dei passaggi parlamentari nei quali si sono registrati importanti modifiche rispetto al testo originario presentato dal Governo. Sull'importanza e sul senso della misura principale contenuta nel decreto, fortemente contestata dall'opposizione, che consente il concorso straordinario dello Stato per il ripiano dei disavanzi dei servizi sanitari regionali registrati nel periodo 2001-2005, per un ammontare di tre miliardi di euro per il 2007, ho già avuto modo di soffermarmi durante le dichiarazioni rese nella prima lettura del provvedimento. Vorrei semplicemente ribadire che nonostante le condivisibili critiche circa la palese incapacità gestionale della spesa sanitaria registratasi in alcune Regioni fino a questo momento, il concorso statale risulta essere indispensabile al fine del successo della seria politica dei piani di rientro dai *deficit* strutturali sottoscritti dalle Regioni. Ciò in ossequio al principio fondamentale del federalismo solidale. Oggi vorrei focalizzare la mia attenzione sulle importantissime modifiche che hanno trovato compiuta sintesi nel testo sul quale il Governo ha posto la fiducia alla Camera. Per quanto attiene alla completa abolizione dei *ticket* sulla diagnostica, la misura, fortemente attesa, dimostra un alto senso di responsabilità del Governo e del Parlamento nei confronti dei cittadini. È con particolare soddisfazione che registro, poi, l'accoglimento di rilievi mossi dall'Udeur in merito alla copertura di tale misura per la quale, in un primo momento, si voleva attingere iniquamente, tra gli altri, al fondo per le famiglie. Viene poi correttamente eliminata la moratoria di 12 mesi dei pignoramenti delle somme dei decreti ingiuntivi contro le aziende sanitarie che non pagano i fornitori. Tale misura, che aveva da subito registrato la contrarietà dell'Udeur, sarebbe stata molto pericolosa sia dal punto di vista sociale che economico, poiché le conseguenze sarebbero ricadute sui cittadini e sulle imprese. Da ultimo, ma non per importanza, le previsioni di di un maggiore coinvolgimento del Parlamento, che riceverà annualmente una relazione sullo stato dei debiti; della trasmissione alle competenti Commissioni di Camera e Senato

ma perché oggi qui non stiamo parlando di Sanità - riguardo alla quale la Lega è assolutamente d'accordo che debba essere garantita a tutti i cittadini - e nemmeno di *ticket*, visto che li avete messi voi e poi li avete tolti su sollecitazione nostra; quindi non è questa la questione. Oggi si sta parlando di amministrazione della "cosa pubblica"

gestisce male, per cui vi sono Regioni, come la Lombardia, il Veneto, il Piemonte, la Puglia, che o fanno un bilancio direttamente a zero oppure si arrangiano da soli a coprire eventuali disavanzi, e abbiamo Regioni che invece sperperano, spendono soldi in cose assolutamente inutili, sono incapaci di gestire i propri amministratori e i propri responsabili sanitari, creano buchi nella Sanità della loro Regione e alla fini questi buchi vengono coperti dai cittadini delle Regioni che già si pagano la propria sanità. È una situazione assolutamente inaccettabile. Almeno ci fosse stato un minimo di messaggio di moralizzazione per il futuro: abbiamo presentato emendamenti per dire che almeno andiamo a punire gli amministratori che fanno queste cose, invece nemmeno questo, copriamo e basta. Nel momento in cui state già ammazzando la metà del Paese che lavora con la chiusura dei negozi dopo tre scontrini mancati, con gli studi di settore che arrivano a far pagare il 200 per cento sugli utili che non esistono alle aziende, permettete ad amministratori che fanno buchi di miliardi di euro di continuare ad amministrare esattamente come prima. L'economia - noi che amministriamo il Paese dovremmo saperlo bene - è una gioco a somma zero: se qualcuno perde qualcun'altro deve ripianare la perdita. Quindi, non esiste il diritto alla sanità delle famiglie e dei cittadini e basta, ma il dovere di tutto il Paese di pagarsi la propria sanità. Voi oggi avete sancito il principio che c'è chi paga e c'è chi sperpera, e chi paga lo fa anche per chi sperpera.

i *ticket* ai cittadini. Ricordo alla signora Turco che la Lombardia ha chiuso la propria sanità in pareggio, che i cittadini lombardi pagano le tasse per la sanità e per il resto e dovrebbero essere presi ad esempio, invece di andare ad indicare al resto del Paese la via della furbizia, per cui si sperpera, si spende, tanto alla fine ci sono i contribuenti padani che pagano per tutti. Questo non va bene. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione i vari interventi che si sono succeduti in quest'Aula sul decreto-legge 20 marzo 2007, n. 23, recante disposizioni urgenti non per il risanamento dei conti, che è un'altra cosa rispetto all'intervento del senatore di maggioranza che voleva sostenere questa tesi, quanto piuttosto per il ripiano selettivo dei disavanzi pregressi nel settore sanitario con riferimento all'abolizione della quota fissa sulla ricetta per la prescrizione di assistenza specialistica ambulatoriale, che questo Governo e la maggioranza di centro-sinistra avevano posto. è inoltre presa in considerazione la cancellazione dal provvedimento del blocco per 12 mesi dei pignoramenti da parte dei creditori del servizio sanitario nazionale nelle Regioni con i conti in rosso nel 2005, che avrebbe costretto le stesse, qualora non fosse stato modificato, a chiudere i battenti e a licenziare i lavoratori. Esistevano profili di incompatibilità rispetto alla disciplina comunitaria in materia di transazioni che avrebbero sicuramente determinato l'attivazione di procedure di infrazione della direttiva 2003/35 relativa alla lotta contro ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e conseguentemente riflessi finanziari non previsti in termini di sanzioni e spese. Si tratta dell'ennesimo intervento legislativo adottato nel corso degli ultimi anni per far fronte al ricorrente problema dello sforamento da parte delle Regioni dei limiti di spesa per il finanziamento del servizio sanitario nazionale con il quale si interviene mediante un ripiano di tre miliardi di euro, dichiarato selettivo sui disavanzi regionali nel settore sanitario per il periodo 2001-2005. ogni caso di un provvedimento che viola il principio di uguaglianza delle Regioni, che attua una palese discriminazione, che premia quelle più inefficienti e meno capaci dividendole in Regioni amiche e Regioni più amiche. A proposito della selettività ed ingerenza nelle competenze regionali, risulta che le due Giunte regionali della Lombardia e del Veneto, in data 28 marzo 2007, abbiano deliberato di impugnare il decreto-legge in esame promuovendo il giudizio di legittimità innanzi alla Corte costituzionale, con riferimento sia al rispetto delle competenze legislative definite, sia a quello di altri princìpi costituzionali. ricordi anche che la stessa Regione Veneto ha addirittura disposto, intervenendo con risorse proprie e prima che la stessa Camera intervenisse con l'abolizione del *ticket*, l'eliminazione di questa tassa iniqua. Si è violato il principio della ripartizione della potestà legislativa che, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, attribuisce compiti alle Regioni e riserva allo Stato una competenza esclusiva solo sulla definizione dei LEA, i cosiddetti livelli essenziali di assistenza, ma non interviene su quello dell'organizzazione ed erogazione e nemmeno sullo svolgimento di badante nei confronti di quelle Regioni che hanno i conti in rosso. Ora, è difficile, pur senza fare ricorso alla dietrologia, non supporre che la sanità sia stata considerata da queste Regioni un formidabile strumento clientelare usato non tanto per governare la sanità quanto piuttosto i dipendenti e i loro voti. vorrebbe anche capire se, in presenza di una evidente discriminazione, persistente sia tra quelle Regioni che hanno accumulato disavanzi nel periodo 2002-2005 e ammesse al finanziamento, oltre che tra quelle che hanno adottato comportamenti virtuosi, non si sia violato anche il principio di eguaglianza o se possa essere considerato come buon andamento della pubblica amministrazione il sanare inefficienze di alcune Regioni disincentivando e demotivando le altre, che invece hannoadottato comportamenti virtuosi. Torno a sottolineare che con questo provvedimento si penalizzano le Regioni che non hanno i conti in rosso, ma soprattutto i cittadini residenti nelle suddette Regioni, che hanno pagato più tasse per riequilibrare i debiti del servizio sanitario nazionale e che da adesso potranno usufruire per di più di minori risorse statali mentre contestualmente accade che si premiano le Regioni meno virtuose, che ancora una volta allegramente possono contare su un ripiano *a* *posteriori* degli sfondamenti di spesa prodotti. Una delle modifiche significative apportate nell'*iter* alla Camera a questo provvedimento è stata, oltre all'eliminazione dell'impignorabilità delle ditte creditrici verso le aziende, l'abolizione per il 2007 del *ticket* di 10 euro sulle prestazioni specialistiche. Ricordo che gravissime perplessità erano state suscitate dalle iniziali modalità individuate per la copertura degli oneri derivanti dalla precedente diminuzione apportata in quest'Aula. Una copertura attuata, dopo la remissione all'Aula da parte del Governo, mediante la riduzione dei fondi destinati ai Paesi in via di sviluppo, fondi destinati alla ricerca nel settore della salute, al Fondo delle politiche per la famiglia, che già ne aveva pochi, al Fondo per le non autosufficienze, che non ha alcuna risorsa, al Fondo per le politiche giovanili, al Fondo unico per lo spettacolo. La copertura, successivamente cambiata alla Camera, deriva per la maggior parte dell'onere dal Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Riflettendo su quanto accaduto in questi anni, non possiamo non rilevare che con la cosiddetta riforma aziendale delle ASL e degli ospedali, la cosiddetta riforma Bindi, introdotta dall'allora Ministro della sanità, la situazione sanitaria non sia affatto migliorata in questo Paese: si è passati da una gestione definita da molti baronale, cioè in mano ai medici, ad una gestione aziendale e manageriale, che ha, tuttavia, aggravato ancora di più i problemi esistenti. Una gestione - vale la pena sottolinearlo - che continua a subire costantemente l'ingerenza politica in tutte le Regioni, sia quelle virtuose, sia quelle meno, e non impedisce l'eliminazione degli sprechi nelle strutture esistenti. Troppo spesso accade che i cosiddetti *manager* prendano decisioni che non favoriscono la buona amministrazione della sanità, ma soltanto interessi particolari. Su questo, fino ad oggi, il ministro Turco non è andata al di là delle buone intenzioni e delle molte parole: ha parlato della casa della salute, dove si dovevano incontrare le varie rappresentanze sindacali, quelle sanitarie e quelle professionali, al fine di discutere e programmare il cosiddetto patto per la salute. Parole. Al di là delle parole, però, poco, troppo poco è stato fatto. La sanità continua a sfuggire al controllo e alla responsabilità e si mostra sempre più incapace di superare le lungaggini delle liste d'attesa, imperdonabili, e le disfunzioni organizzative. Resta così il sospetto che i supposti piani di rientro che sono stati inseriti dal decreto-legge in oggetto finiscano con l'essere non tanto dei piani virtuosi di risanamento, ma semplicemente dei piani economici, dove attraverso le economie

Concludendo, non ci convince affatto la politica del cosiddetto vitello grasso, che viene sistematicamente offerto ad alcune Regioni e che evita sapientemente di ospitare a tavola altri commensali, quelli cioè che hanno dimostrato maggiore serietà e responsabilità, oltre che oculatezza nella gestione delle risorse. Si tratta di una politica profondamente iniqua e diseducativa; sappiamo bene che i malati sono incolpevoli, ma non lo sono sicuramente gli amministratori e i dirigenti. Le sanatorie per gli enti locali che hanno sforato i patti di stabilità hanno un che di usuale e ripetitivo. Sta vigendo, purtroppo, nella sanità, ma anche per l'emergenza rifiuti in Campania, la stessa Regione che qui figura come beneficiaria dei fondi in oggetto, l'incentivazione di comportamenti irresponsabili. È per tale ragione e per quelle che abbiamo precedentemente affermato nel corso del dibattito che l'UDC conferma, anche in questa terza lettura, il voto contrario del proprio Gruppo.

di ironizzare, guardate dentro casa vostra e capite che certe battaglie sono comuni. Quel *ticket* era un'idiozia. Lo avete riconosciuto, avete fatto bene a toglierlo, però imparate che il dialogo serve non solo a noi, ma anche e prima di tutto a voi.

che nel piano di ristrutturazione del Servizio sanitario regionale è prevista anche la cancellazione come struttura ospedaliera dell'ospedale San Giacomo. Ricordo che nel 1999 al San Giacomo

sulla richiesta dell'opposizione di abolire i *ticket* sulla diagnostica. Si è verificato anche uno scontro alla Camera

Signor Presidente, una politica sanitaria efficace dovrebbe assumere una visione lungimirante, evitare il prevalere di logiche economicistiche, ma, nel contempo, dovrebbe essere in grado di individuare le aree di disfunzione e di non appropriatezza sulle quali è possibile recuperare risorse da riconvertire sulle aree a maggiore impatto strategico per la salute collettiva e per il miglioramento del sistema assistenziale. In altre parole, una politica sanitaria oculata deve indirizzarsi verso logiche di razionalizzazione e non di razionamento. È per tale ragione che il Governo ha ritenuto indispensabile provvedere con questo decreto‑legge a varare provvedimenti urgenti e incisivi per superare la situazione debitoria di alcune Regioni italiane. Un'eredità pesante che non consente più ad alcune aree del Paese di provare ad inverare i princìpi e i valori fondanti del nostro Servizio sanitario nazionale, così come prefigurato dall'articolo 32 della Costituzione: la salute come un diritto da promuovere e tutelare e non come bene da negoziare, l'equità e l'universalismo intesi come pari opportunità di accesso e di fruizione dei servizi sanitari da parte di tutti i cittadini e le cittadine presenti a qualunque titolo sul territorio nazionale e in qualunque Regione italiana. Per questo oggi, pur nella necessità di ripianare *deficit* che hanno raggiunto le cifre e le situazioni debitorie di cui abbiamo parlato, si decide di invertire una tendenza e, a fronte del concorso economico selettivo dello Stato, si richiede alle Regioni di operare tagli di spesa anche su aree extrasanitarie, consci del fatto che gli effetti di una politica di tagli sanitari indiscriminati tenderebbero a rendersi progressivamente evidenti su tutta la comunità, in particolare sulle fasce socialmente più deboli. Il decreto assume quindi la necessità che lo Stato e le Regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare strategie condivise al fine di superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilità e di promozione di una sempre maggiore qualità dei servizi. Rifondazione Comunista condivide il merito di questo provvedimento che affronta in particolare due questioni: la prima è lo stanziamento per il ripiano dei disavanzi sanitari delle Regioni in grave stato debitorio del periodo 2001-2005. Vorrei ricordare - soprattutto ai colleghi dell'opposizione - che la stessa misura è stata già adottata per ben due volte e per un importo complessivo di 4 miliardi di euro anche nella precedente legislatura, ma, a differenza di questa volta, senza che il Governo ponesse alle Regioni, i cui debiti ripianava, alcun vincolo e senza alcuna misura strutturale che potesse invertire la tendenza al passivo. Questo finanziamento, invece, si rende necessario per garantire a tutti cittadini il diritto universale alla salute indipendentemente dal luogo in cui vivono. Senza di esso, infatti, alcune Regioni sarebbero costrette a ridurre il livello dei servizi sanitari, a chiudere ospedali e reparti, a smantellare servizi di assistenza territoriale, a cancellare programmi di prevenzione. Credo che nessun collega qui dentro, nemmeno i colleghi della Lega che tanto di solito lavorano per il federalismo, possa accettare una simile prospettiva. Tutti noi sappiamo che la situazione debitoria deriva da due cause. In primo luogo, dal sotto finanziamento della spesa sanitaria; non è vero infatti che in Italia si spende troppo per la sanità, anzi, si spende poco in rapporto agli altri principali Paesi europei.

che alla Camera avevamo presentato in questo e in diversi altri provvedimenti, riguarda tutti i cittadini italiani e consiste nell'abolizione del *ticket* di 10 euro sulle ricette per le prestazioni specialistiche e ambulatoriali. ci riempie di soddisfazione perché segna il successo di un'azione che Rifondazione Comunista ha sempre condotto contro i *ticket* e, nel caso specifico, fin da quando essi furono introdotti nell'ultima legge finanziaria. Già da allora Rifondazione Comunista si è battuta, spesso da sola, contro questa decisione e in finanziaria non siamo stati ascoltati. I *ticket* non possono essere considerati uno strumento di controllo della spesa sanitaria e ancora meno un modo per incassare risorse, ma sono una misura odiosa e ingiusta perché colpisce il cittadino proprio nel momento del massimo bisogno, quando è malato, e colpisce di più le persone e le famiglie meno abbienti, per le quali anche poche decine di euro possono produrre difficoltà economiche e costringere a sofferenze e rinunce. Il diritto alla salute deve essere assicurato a tutti, ricchi e poveri, italiani e stranieri, e per tale motivo deve essere garantito dalla sanità pubblica e finanziato attraverso la fiscalità generale e progressiva in forma solidaristica, in modo che chi ha di più contribuisca di più a garantire la vita e la salute di tutti. Siamo contenti che oggi anche il Governo abbia riconosciuto l'inutilità e l'ingiustizia del balzello del *ticket* sulle ricette. L'abolizione del *ticket* è un esempio di ciò che concretamente intendiamo quando parliamo di utilizzare le risorse derivanti dal maggior gettito tributario per una grande operazione di risarcimento sociale e di redistribuzione del reddito. Grazie all'azione fin qui condotta, due delle tre gravi emergenze lasciate in eredità dal Governo Berlusconi, quella economica e quella finanziaria, sono state ridimensionate. È questo un grande merito del Governo e della maggioranza. Ma oggi, se consideriamo le condizioni sociali del Paese, ci accorgiamo che non sono molto diverse da quelle disastrose che abbiamo ereditato da cinque anni di Governo Berlusconi. Chi vive di pensioni e di salari, chi è disoccupato, chi è immigrato, insomma, la grande maggioranza della popolazione che produce la ricchezza del Paese, oggi non sta meglio di un anno fa. La diseguaglianza nella distribuzione del reddito e della ricchezza, purtroppo è ancora enorme. Riteniamo quindi giusto e indispensabile che le risorse siano utilizzate per ridurre quella diseguaglianza, per migliorare le condizioni di vita delle fasce più deboli. Come dimostra la vicenda del *ticket*, oggi finalmente abolito, le proposte di Rifondazione Comunista non nascono da una visione ideologica ed estremistica, né tantomeno sono finalizzate a creare instabilità e difficoltà nell'azione del Governo, anzi, è vero l'esatto contrario. Quando chiediamo misure di redistribuzione, con proposte concrete e praticabili, come questa volta, intendiamo collaborare con il Governo e spingerlo a migliorare la propria azione e ad estendere il proprio consenso.

colleghe e colleghi, voglio distinguere nella mia dichiarazione di voto alcune considerazione sulla parte del provvedimento che riguarda

tutte le Regioni in difficoltà. Infatti, il fondo sanitario stanziato dall'ultima finanziaria, nonostante abbia riportato un incremento rispetto all'anno precedente, registra una situazione di forte criticità

del problema sanitario, esattamente equiparabile a quello previdenziale. Lì c'è una forbice che prima o poi si incontrerà e porterà chiaramente al dissesto non solo di alcune Regioni ma di tutto il sistema sanitario nazionale. La conseguenza è che il provvedimento

altre amministrazioni regionali non lo fanno. Alla fine il Governo vanifica una politica di rigore realizzata in questi ultimi dieci anni: ricordo a tutti il concetto proposto dal sottosegretario Giarda per cui chi rompe paga, in buona sostanza il patto tra le Regioni ed il Governo, nel tentativo di mantenere la spesa sanitaria sotto controllo. Questo provvedimento oltretutto presenta evidenti elementi di incostituzionalità, tant'è vero che alcune Regioni hanno già fatto ricorso alla Corte costituzionale, ed ha, come detto, il grossissimo difetto di non risolvere, se non attraverso una misura tampone, nessun tipo di criticità che nel sottofondo si vede.

dovranno comunque ricorrere alla tassazione regionale di IRPEF e IRAP per coprire, attraverso il piano di rientro, una parte di disavanzo che non viene coperto, se non in minima parte, dallo stanziamento di questo provvedimento che è di 3 miliardi di euro,

che esiste ancora il *ticket* del pronto soccorso, di cui richiediamo con forza l'abolizione. Per queste ragioni e per evitare che ci siano elementi che possano essere interpretati in senso contraddittorio della nostra posizione, ci asterremo definendo in modo chiaro che siamo contrari alla prima parte del provvedimento e favorevoli alla seconda. Ma poiché il provvedimento è uno solo, Forza Italia si asterrà. *(Ulivo)*. Esporrò molto brevemente le ragioni per cui il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore del provvedimento. E lo farò proprio per riuscire a rispettare tempi brevi, cercando di rispondere alle quattro questioni principali poste nel dibattito. Già altri colleghi, intervenendo in discussione generale, lo hanno fatto. Io sintetizzerò le opinioni già espresse.

come un elemento della strategia del Governo per affrontare in modo definitivo il problema della spesa sanitaria. Ricordo i tre punti contenuti nella legge finanziaria: certezza delle risorse per un triennio; un triennio; responsabilità delle Regioni chiamate ad affrontare con risorse proprie lo scostamento dai risultati di efficienza concordati; necessità di affrontare il problema del rientro per le Regioni che presentano forti disavanzi.

con riferimento agli interessi dell'intero sistema. Ce lo ha ricordato molto bene il Ministro nel suo intervento in prima lettura, che condivido. Se non risolviamo il problema di Regioni il cui sistema sanitario rischia di esplodere per un eccesso di debito rischiamo di minare

con l'alimentare un mostruoso circuito negativo che moltiplica all'infinito il debito sanitario. Era quindi necessario e si inserisce dentro una strategia: non è un provvedimento tampone. La seconda critica fatta da molti colleghi intervenuti è la seguente: si tratta di un regalo a qualche Regione. Anche qui, è già stato ricordato in qualche intervento, ci troviamo in presenza di un meccanismo molto diverso rispetto a quello realizzato in passato anche dal precedente Governo di centro-destra. Si prevede un intervento a ripiano del disavanzo, ma si tratta di un intervento di ripiano vincolato al rispetto di impegni molto stringenti. Ci sono impegni alla predisposizione, all'approvazione e alla firma di piani di rientro da parte delle Regioni fortemente indebitate. Ci è stato comunicato quasi tutti questi accordi per i piani di rientro sono stati firmati dalle Regioni interessate e sono previste misure di accompagnamento da parte del Governo.

La terza critica che è stata rivolta è quella secondo la quale ci troveremmo in presenza di un intervento a carattere diseducativo.

Riconosco che questo è un problema su cui dobbiamo riflettere e che sarebbe stato opportuno accompagnare questo provvedimento introducendo anche un meccanismo premiale per le Regioni virtuose. È un problema che consideriamo aperto e che intendiamo affrontare nel prossimo futuro; si tratta di una riflessione che condividiamo debba essere svolta. La quarta critica rivolta, molto puntuale, è relativa alla questione delle coperture.

Ricordo soltanto che il meccanismo di copertura indicato dal Governo, pur se problematico, garantisce garantisce il bilancio dello Stato, perché ci troviamo in presenza di un fondo che ha la necessaria capienza e le cui necessità di utilizzo sono collocate nel tempo in una posizione tale

Le preoccupazioni che anche la Commissione bilancio ha espresso in ordine ai meccanismi di copertura sono superate dalla garanzia che il Governo ci ha dato; noi stessi abbiamo verificato che il meccanismo di copertura, pur se problematico, funziona.

esame - e lo faremo - noi convintamente richiamiamo gli italiani al fatto che interveniamo abolendo i *ticket* e avviando un tempo diverso per quanto riguarda il finanziamento della spesa sanitaria del nostro Paese.

Presidente, il senatore Stefani ha prima articolato le motivazioni per le quali riteniamo assolutamente necessario porre all'ordine del giorno anche questa materia, atteso che in Commissione c'è stato un vivace dibattito anche sulla questione relativa all'opportunità di riprendere in esame, almeno a livello di ricerca, le questioni sull'energia nucleare. Ora sta venendo avanti, anche da parte dei Verdi (sto parlando dell'ambiente internazionale dei Verdi), la consapevolezza che l'unico sistema per poter combattere l'effetto serra sia quanto

che ci fosse una sostanziale unanimità da parte dei Gruppi perché l'argomento potesse essere inserito all'ordine del giorno ed eventualmente iniziata la relazione se mi è stato riferito in maniera diversa). Dico questo perché, se la richiesta venisse accolta da parte dell'Aula, senza particolari procedure, non sarebbe necessaria una sequenza di votazioni elettroniche che porterebbe sicuramente, per almeno quattro volte, alla mancanza del numero legale.

perché la Presidenza del Senato e la Conferenza dei Capigruppo hanno stabilito che il termine per la presentazione degli emendamenti a questo provvedimento scade il giorno 24. 24. Non è possibile che noi incardiniamo e incominciamo l'esame di un provvedimento - la richiesta è anche di votarlo,

termini. Sottoporrei quindi all'attenzione della Presidenza questo elemento di improcedibilità. Signor Presidente, mi rendo poi conto che se la Presidenza non accogliesse questa osservazione, avrebbe di conseguenza ragione il vice presidente Calderoli: mancherà il numero legale. A questo punto, annunzio che noi non concorreremo a che il numero legale ci sia,

la Presidenza si "accanisca" nella riconvocazione ogni venti minuti, perché comunque noi non ci saremo per assicurare il numero legale. Ciò mi pare doveroso nei confronti dei colleghi dell'opposizione e anche del vice presidente Calderoli, verso il quale non ci sentiremmo di fare un dispetto e al quale comunico come stanno le cose con molta lealtà e serenità.

definitivi la possibilità di presentare emendamenti al provvedimento, ma è altrettanto vero che è possibile - ancorché non procedere ad alcuna votazione procedere però alla discussione del provvedimento medesimo. Quindi, in teoria c'è una legittimità formale della richiesta del collega Calderoli.

votazione. Noi intendiamo proporre all'Assemblea - non vedo proprio motivi contrari, se non eventuali pressioni di Confindustria - di incardinare il provvedimento per essere certi che, alla ripresa dei lavori, il provvedimento medesimo venga affrontato,

Lasciamo stare le strumentalità; qui ci sono le richieste formali di diversi colleghi rispetto alle quali gli altri colleghi si esprimono a favore o contro: non c'è alcuna strumentalità da parte di nessuno.

sono a chiederle l'aggiunta all'ordine del giorno, ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento del Senato, del provvedimento A.S 691 "Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie del 2003/54/CE,

finestra"). Ricordo ai colleghi che domani il Parlamento sarà riunito in seduta comune per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale, alle ore 10. Ricordo che i colleghi senatori voteranno per primi.

qualche settimana fa, quando ci fu tutto quel movimento sulla politica estera che ricordiamo tutti. Essendo successe esattamente le cose che chiedevamo e che i rappresentanti della sinistra non volevano (in cambio del voto favorevole che poi c'è stato), ci piacerebbe capire in base a cosa si sia proceduto a questo rafforzamento della nostra presenza nell'area, in palese contrasto con quanto deciso anche in quest'Aula qualche settimana fa. Quindi, le chiederei di inviare richiesta al Ministro...